Onorevoli colleghi, è di poche ore fa la notizia dei drammatici attentati terroristici che hanno colpito la città di Bruxelles. Le informazioni giunte questa mattina riferiscono di esplosioni nella sala partenze dell'aeroporto della capitale belga e di altre deflagrazioni all'interno della metropolitana, vicino alle sedi delle istituzioni europee. Sono passati poco più di quattro mesi dagli attentati di Parigi e nuovamente ci troviamo a fronteggiare efferati atti di violenza e la lucida follia omicida di chi rifiuta i fondamenti della convivenza civile. Oltre alla loro tragicità, questi attentati assumono anche una valenza simbolica, poiché colpire Bruxelles significa colpire l'Europa e i suoi valori; è quindi necessario che la risposta sia corale e unitaria in un quadro di fermezza. La Presidenza esprime ai parenti delle vittime e alla popolazione del Belgio i sentimenti di cordoglio e di solidarietà del Senato italiano. Invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio.

Come è noto, sette studentesse italiane hanno perso la vita in un tremendo incidente stradale che ha provocato complessivamente 13 morti e 34 feriti, di cui alcuni in condizioni molto gravi. Francesca Bonello, Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini, Serena Saracino, Elisa Scarascia Mugnozza, Elisa Valent, sono i nomi delle nostre ragazze che si trovavano in Spagna nell'ambito del progetto Erasmus. È veramente difficile rassegnarsi all'idea di come i sogni e le aspettative di queste giovani studentesse, partite per vivere un'importate occasione di crescita e di formazione umana e culturale,

Serena, Elisa ed Elisa va l'abbraccio di tutti noi. Invito anche in questo caso l'Assembla a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento.

siamo qui oggi perché, alla fine, la riforma del terzo settore, uscita dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 2014 e da più di un anno all'esame delle Camere, è approdata nell'Aula del Senato, cioè dopo un anno esatto, nonostante il Governo avesse preso l'impegno di far approvare la legge delega entro il 2015. Il testo, approvato dalla Camera il 13 aprile scorso, è arrivato al Senato, che ha iniziato a discuterlo in Commissione affari costituzionali È doveroso ricordare che con 5 milioni di volontari, 12.000 cooperative sociali, almeno 800.000 occupati, oltre 300.000 istituzioni attive, il mondo del *no profit* rappresenta circa il 4 per cento del PIL. Pertanto, anche sotto il profilo occupazionale, si attendeva una legge capace di disciplinare meglio il terzo settore da circa venti anni. Il concetto di terzo settore - è bene ricordarlo - deriva dalla considerazione dell'esistenza nel sistema economico e sociale di un primo settore rappresentato dallo Stato e di un secondo costituito dal mercato. Si identifica, di solito, con l'insieme di attività produttive che non rientrano né nella sfera dell'impresa capitalistica tradizionale né in quella delle amministrazioni pubbliche. Insomma, il terzo settore è costituito da tutte tutte quelle realtà che, all'interno del nostro sistema socio-economico, si collocano a metà tra Stato e mercato; ne integrano le funzioni, coprendo spazi strategici per le istituzioni e per la vita della stessa della democrazia. Diverse per struttura organizzativa (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati) e per natura giuridica (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, società di mutuo soccorso imprese sociali e ONLUS), le realtà del terzo settore hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali, tra le quali l'assenza di scopo di lucro, che si si traduce nell'obbligo di reinvestire gli eventuali utili nelle attività istituzionali e nella natura giuridica privata. Operano in numerosi settori quali l'assistenza sociali, la sanità, la cultura, lo sport, la cooperazione internazionale, l'istruzione e la ricerca, l'ambiente, lo sviluppo economico e sociale, la promozione e la formazione religiosa, la promozione del volontariato. Siamo ragionevolmente critici su questo disegno di legge. Infatti, come sempre e più spesso accade, ciò che viene dichiarato ad alta voce dalla maggioranza non corrisponde poi al contenuto dei testi proposti.

Dopo un *iter* incerto, che in alcuni momenti ha fatto temere l'accantonamento del provvedimento per incapacità di sostenerne l'onere economico, la scorsa settimana si sono chiusi a sorpresa i lavori in Commissione, ma non prima che il Governo presentasse un alquanto dubbio emendamento per l'istituzione della Fondazione Italia sociale, puntualmente ribattezzata l'IRI del sociale. Fortunatamente le opposizioni - in particolare, noi Conservatori e Riformisti - hanno tenuto a rimarcare le perplessità dettate dall'istituzione di tale organismo, anche attraverso un'attività emendativa incisiva,

Si parla di un servizio civile universale, ma non c'è questa universalità perché mancano le risorse e i bandi non vengono pubblicati, come è stato ricordato. Si danno una Si danno una timida impostazione e un timido avallo a un nuovo tipo di impresa sociale ma, nel contempo, ci si rifiuta di applicare interamente quanto prevede la normativa per le *start-up* a vocazione sociale in termini di fiscalità di favore per chi investe - cittadini o imprese - e si dice che costerebbe troppo (qualche punto percentuale rispetto alla normale fiscalità di favore, a vantaggio delle *start-up* innovative, per così dire, semplici). Per non parlare degli altri profili lasciati inesorabilmente da parte dal disegno di legge in esame, come il riconoscimento della figura professionale dei *caregiver* familiari (cioè volontari che si prendono cura di persone care in condizioni di non autosufficienza), che ad oggi ancora non esiste in Italia. Il 13 gennaio 1986 il Parlamento europeo ha invece approvato ha invece approvato una risoluzione che ha individuato l'importanza del lavoro non remunerato delle donne. A livello europeo, la legislazione di molti Paesi prevede specifiche tutele per i *caregiver* familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene soprattutto in Francia, Spagna e Gran Bretagna. Anche su questo punto il Gruppo parlamentare cui appartengo ha presentato un emendamento, le cui finalità sono state tuttavia disattese. Da questo punto di vista, il provvedimento in esame è veramente una buona occasione sciupata.

Il Governo ha presentato l'ennesima delega a se stesso per riformare un settore in cui si possono nascondere interessi privatistici utilizzando le agevolazioni, fiscali e non, riservate alle imprese che si occupano di solidarietà. Una delle modifiche intervenute nel testo riguarda la cancellazione del termine per la presentazione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere per l'espressione del parere che - ricordiamo - non è vincolante. In base all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega devono essere compensati all'interno della delega stessa. Siccome vi siete resi conto che l'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali comporterà ulteriori oneri per l'erario e quindi maggiori spese per lo Stato, avete modificato questa parte inserendo

o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Non contenti di questo giochino economico-contabile, avete dato un'ulteriore delega al Presidente del Consiglio per individuare ed aggiornare i settori e le attività riferibili al terzo settore, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Anche in questo caso, però, il parere non sarà vincolante. vincolante. In apparenza, quindi, cercate la condivisione e l'indirizzo del Parlamento, ma in realtà state trasportando anche questo settore sotto l'egemonia del Presidente del Consiglio. Che dire poi dell'emendamento del Governo per l'istituzione della fondazione Italia sociale? Casualmente la prima versione dell'emendamento indicava pure la sede legale di tale fondazione

che però manca della linea alta velocità tra Arezzo e Firenze e quindi è sempre in ritardo? Questo Governo è un insieme di conflitti e sospetti. Ricordo a titolo informativo che è di pochi giorni fa l'apertura delle indagini per bancarotta fraudolenta verso tutto il consiglio di amministrazione della Banca Etruria, che coinvolge anche il padre della ministra Boschi. Tutto ciò che l'Esecutivo in carica ha fatto fino ad oggi conferma la sua negligenza e incompetenza, mettendo a rischio l'equilibrio del Paese. Quale delega potremmo mai dare a questa squadra di Governo? Al massimo quella per la riforma della disinformazione, che abilmente sta portando avanti a danno di tutti i cittadini.

che l'impegno del Governo sul provvedimento in esame sia stato pressante e, come sempre accade con l'Esecutivo in carica, ad una corretta volontà di affrontare e mettere ordine in un settore importante, seguono risultati risibili. Era già successo con la debole riforma sulla scuola, che con un po' più di coraggio si sarebbe potuta trasformare in una buona riforma, con la riforma costituzionale, che aveva qualche aspetto positivo, naufragato poi in un mare di contraddizioni ed errori; era successo con il *jobs act*, che non ha avuto la capacità di affrontare veramente i problemi del mondo del lavoro, malgrado le buone intenzioni e i *tweet* sbandierati dal nostro Primo Ministro. Anche il tentativo di mettere ordine nel terzo settore, dopo che abbiamo vissuto anni di impetuoso sviluppo,

che ne aveva capito non solo la grande potenzialità economica, ma il profondo valore sociale. Il luogo della vera sussidiarietà, dell'impegno verso i più deboli, della corretta sostituzione di aiuti statali e statalisti con iniziative liberali e non impegnative per le risorse comuni: questo era ed è per noi il ritratto ideale del terzo settore, indispensabile soprattutto in questa epoca in cui la coesione sociale si sta indebolendo di fronte a crisi economiche epocali, a scenari di guerra, terrorismo ed immigrazione selvaggia. Non solo. È anche la dimostrazione di quanto possano essere efficaci politiche fiscali mirate a permettere al singolo cittadino di intervenire in aiuto di chi si occupa degli altri. Stiamo parlando di 5 milioni circa di volontari, 12.000 cooperative sociali, più di 800.000 occupati: un impatto del 4 per cento sul PIL. Tutto questo meritava sicuramente tempi più veloci, attenzione particolare e approfondimenti migliori. Si è scelta invece la strada della delega sostanzialmente in bianco, che si limita a indicare la necessità di riordino e revisione delle discipline, senza prevedere la qualità e le linee guida di questo riordino, peraltro necessario. Sembra, insomma, di intuire un'azione di semplice limatura burocratica, di miglioramento dell'esistente, senza che si riesca a disegnare la strada del futuro, senza provare neanche a comprendere quali saranno le tendenze per lo sviluppo del settore. Come sempre, un provvedimento povero, senza coraggio, senza prospettive. Ciò non toglie che ci siano degli elementi parzialmente positivi. Sperando che non rimangano lettera morta, sono comunque lodevoli l'intenzione di misurare l'efficacia delle azioni di chi opera nel terzo settore, e la volontà di aumentare la trasparenza e quindi di diminuire il rischio che si ripetano scandali come quello di Roma Capitale, tutto interno al terzo settore. Anche su quest'ultimo aspetto sarebbe stato necessario un maggiore coraggio, una delega più precisa e puntuale che intervenisse sui meccanismi di distribuzione degli appalti e dei fondi, ma comunque è da valutare positivamente l'intenzione, in questo campo, del provvedimento. Starà a noi vigilare affinché queste deboli luci presenti nella legge delega non vengano poi spente durante l'attuazione delle deleghe. C'è infine un ultimo punto che voglio prendere in considerazione. Il relatore, ad un certo punto dei lavori in Commissione, ha presentato un emendamento che avrebbe stravolto non solo il senso del provvedimento, ma l'intera esistenza del mondo *no profit* in Italia. Si prevedeva infatti la nascita di una nuova istituzione, la Fondazione Italia sociale, che avrebbe avuto lo scopo di investire fondi (statali e privati), direttamente o in partenariato con altri soggetti, su progetti del terzo settore. Detto in altre e più chiare parole, avrebbe avuto il compito di intermediazione statale e di indirizzo sui fondi che privati o aziende intendono donare alle aziende del terzo settore: come l'hanno chiamata da più parti, insomma, un'IRI del sociale. Bene, grazie all'assoluta contrarietà di tutte le opposizioni, questo emendamento è stato ritirato e riassorbito in un ordine del giorno. Oggi, però, mi sembra di capire, alla luce dello *speech* che abbiamo ascoltato, che questo emendamento, che era

Voglio però affermare la nostra profonda contrarietà a un tentativo goffo e palese di fare intervenire lo Stato in una filiera, quella tra donatori e organizzazioni, che è oggi sul terreno privato. Voglio anzi sottolineare che, dove il terzo settore ha rivelato sacche di corruzione e criminalità, è stato proprio quando interveniva il denaro pubblico, come nei casi di Roma o del CARA di Mineo. Voglio chiudere con una breve considerazione. Avremmo avuto bisogno, in un settore così importante per il nostro Paese, di un provvedimento lungimirante, in grado di guardare avanti, di prevedere i futuri possibili, di ridurre i rischi e aumentarne le possibilità.

il volontariato ha per sua natura e costituzione tipologica una valenza educativa e formativa tuttavia sembra ormai, sempre più spesso, il risvolto opacizzato, poco appariscente, rovesciato di segno, di una società volta esclusivamente al

*b)*, al mondo scolastico e dunque all'aiuto vicendevole e alla collaborazione reciproca. Nel testo si parla, infatti, della «promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche». Ciò va di pari passo con le "magnifiche sorti e progressive" della Buona scuola, laddove fra gli obiettivi formativi prioritari, ai sensi appare esplicitato lo «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace Tutti conosciamo quel bel proverbio africano che sostiene che chi corre da solo va veloce, ma chi corre insieme, con gli altri, va lontano. Purtroppo però il volontariato è chiamato sempre più spesso a surrogare e a tamponare le deficienze dell'organizzazione statale, in moltissimi e in troppi campi: dalla sanità al soccorso alle persone bisognose, dall'istruzione al sostegno ai disabili. Una Repubblica fondata teoricamente sul lavoro forse, primariamente, dovrebbe essere fondata sulla dignità della persona - si basa sempre più sulla buona volontà dei cittadini e sulle strutture e infrastrutture messe in campo dal volontariato. Ora, è un fatto che il volontariato nel suo complesso possa avviare

dobbiamo considerare il contesto nel quale tali concetti risultano espressi. Primo, secondo e terzo; oro, argento e bronzo; primario, secondario e terziario; agricoltura, industria e servizi: fin qui è tutto chiaro, poi cominciano le difficoltà. Possiamo considerare come primo settore l'iniziativa privata, come secondo settore quella pubblica, ma il «terzo settore», colleghi, cos'è? È un'indagine linguistica o una definizione giornalistica, che ha ben poco di giuridico? È un ircocervo, ovvero un'iniziativa privata, ma senza scopo di lucro? un abito ben abbottonato dietro il quale nascondersi, o nascondere i propri interessi? Il timore, purtroppo fondato e manifestato praticamente *in toto* dal mondo del volontariato, in merito alla nuova disciplina del terzo settore, millantata e promessa nel disegno di legge in esame, è che la riforma prenda una piega diversa da quella dichiarata e auspicata. In effetti sembrerebbe che non si stia tenendo conto quanto si dovrebbe delle priorità del mondo del volontariato: del principio di sussidiarietà, *in primis*, e della valorizzazione del ruolo del volontariato nella società. Se si pensa che, solo in Umbria, ci sono oltre 100.000 volontari che assistono le cosiddette fasce deboli, ci si può fare un'idea di quanto il volontariato incida sia sulla qualità della vita delle persone, sia sul PIL, dato che vengono così ammortizzati costi altrimenti a carico del sistema sanitario e sociale. Ecco perché è necessario che il variegato universo del volontariato venga adeguatamente riconosciuto, colleghi, e abbia un ruolo ben preciso nel momento in cui vengono compiute le scelte e non venga coinvolto o tantomeno utilizzato a cose fatte. Basti pensare, ad esempio, alla predisposizione del Piano sanitario e del Piano sociale regionale. Le richieste provenienti dal mondo del volontariato da inserire legge di riforma sono innanzitutto quelle di mantenere la gratuità delle prestazioni, poiché il volontariato non vuole diventare impresa. Il mondo del volontariato chiede anche meno burocrazia sul fronte dei controlli, con un *range* minimo di spesa da non considerare reddito ma quale forma di rimborso. Sulla rappresentanza, poi, si chiede di non cancellare gli organi attuali del terzo settore, chiarezza sulla riforma dei centri servizi per il volontariato e la Consulta dei comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato (COGE). Il nostro timore molto più diffuso, invece, è che resti un'ombra, una minaccia che grava sul disegno sfocato di questa riforma: che dietro questa grande macchina si annidi solo il *particulare* di alcuni che - a fronte della tanto decantata «impresa sociale» dal voler essere riconosciuti all'interno del terzo settore possano ricavarne proventi, sgravi e vantaggi. Signor Presidente, tutti noi, senza eccezione alcuna, affermiamo di riconoscere l'importanza del differenziato mondo del terzo settore, ma mi domando se tutti abbiano ben chiaro che cosa significhi realmente, nel bene e nel male, fare volontariato oggi nel nostro Paese; quanto sia defaticante ed impegnativo. Voglio sottolineare la parola «differenziato», perché intanto dovremmo cominciare con il cogliere bene e fino in fondo la pluralità di motivi, sensibilità, modalità operative ed ispirazioni che convivono oggi dentro il terzo settore. Le statistiche ci parlano di PIL generato dal terzo settore, di grandi numeri, di addetti e di volontari, di piccole e grandi associazioni; sulla base della mia esperienza mi sento di dire che questo criterio di valutazione sta stretto al mondo *no profit*. Il metro sul quale una associazione (e in particolare le associazioni che si occupano di temi sociosanitari) misura la propria attività giorno dopo giorno è un altro. Ogni giorno i responsabili delle associazioni si domandano: «Come faccio a rispondere al bisogno, come faccio a dargli voce? Come si fa a sostenere le richieste di servizi che gli enti locali non prestano più e a contrastare il crescente isolamento delle persone più fragili e a tutelarne i diritti? Chi è oggi il mio interlocutore istituzionale? Sono sussidiario alle responsabilità istituzionali o sono chiamato a sostituirle? Come trovare le risorse necessarie?». E poi ancora: «Sono in regola con la normativa?». Tutti questi sono veri e propri incubi quotidiani per ogni volontario impegnato a dirigere un'associazione. C'è un filo storico e culturale che viene da lontano e che unisce la pluralità identitaria tipica del volontariato e di tutto il terzo settore; una cultura che vive da sempre intorno ad alcuni valori essenziali: l'attenzione per le persone in carne ed ossa a partire da quelle più deboli, il non perseguimento di fini di lucro, la solidarietà ed il dono; un dono particolare, che certo può essere anche rappresentato da qualcosa di materiale, ma che soprattutto è dono di sé, del proprio tempo, delle proprie competenze ed abilità, tante o poche che siano. Questo è il senso vero della gratuità e delle finalità *no profit*. La gratuità non è un valore astratto intorno al quale magari alimentare anche qualche filosofica polemica. Se vogliamo parlare di volontariato concreto, quello vero con le sue ombre e le molte luci, quello che opera come può, giorno per giorno, dobbiamo avere ben chiaro che per un associazione sostenere la gratuità vuol dire fare i conti, molto concretamente e molto poco gratuitamente, con le assicurazioni, con i benzinai, con le banche, con le manutenzioni, con gli affitti, con la burocrazia e con una normativa che ormai dice tutto ed il contrario di tutto e che si presta bene come alibi per una certa trasversale politica a non fare niente, a non assumere decisioni e a non assumersi responsabilità (e l'elenco potrebbe essere lunghissimo). Per essere breve, cercherò di focalizzare il mio intervento su pochi punti concreti, punti che, in attesa degli esiti dell'ampia delega prevista nel disegno di legge, auspico possano essere utili spunti di riflessione per chi dovrà tradurre in pratica gli orientamenti di delega presenti nel testo del provvedimento. La legge n. 266 del 1991 rappresentò un importante punto di svolta, anzi di arrivo, per il volontariato e per le istituzioni del nostro Paese. Tale norma riconosceva ufficialmente il ruolo, il senso e l'importanza del mondo del volontariato, un mondo che aveva ed ha ancora al suo centro la cultura della solidarietà, la gratuità,

modalità dei rapporti con le istituzioni, offriva garanzie e poneva vincoli, il tutto in un quadro di chiarezza esemplare. Da quella data ad oggi tante cose sono cambiate e perciò non è strano che sia cambiato anche il volontariato e che il mondo del *no profit* si sia stratificato ed anche eccessivamente diversificato. L'obiettivo di questo disegno di delega, tra le altre questioni, doveva essere - e mi auguro sia tuttora - quello di traghettare quei principi, così ben rappresentati nella nella mutata situazione di oggi. Il volontariato è cresciuto, si è assunto nuove, diffuse responsabilità ed è anche spesso rimasto solo nella sua funzione di *advocacy* di interi settori sociali. Contemporaneamente, le crescenti difficoltà della finanza pubblica hanno indotto gli enti locali a scaricare su di esso nuove funzioni e responsabilità. Per semplicità, credo che possiamo dire che, in qualche modo, è stato anche "dopato". la crisi finanziaria, con la fine di gran parte dei sostegni finanziari, la conseguente chiusura di progetti, iniziative e servizi, il tutto aggravato da una legislazione frammentaria che, anno dopo anno, ha complicato fino all'inverosimile il quadro di riferimento normativo. Dalle convenzioni della legge n. 266 del 1991, chiare e trasparenti, basate su comprovata esperienza operativa, si è giunti oggi a forme di gare inaccettabili, basate, nella sostanza, solo su di una malcelata priorità economica, avviando una specie di competitività anche tra settori diversi dello stesso terzo settore, cioè dando vita a veri e propri mostri amministrativi, culturali e politici. Abbiamo dunque la responsabilità, negli anni, di aver notevolmente contribuito ad inquinare le acque di un mondo che per

bene colpire severamente i furbetti di turno; bene attivare buoni, semplici ed efficaci controlli; ma è impensabile ed ingeneroso generalizzare imponendo a tutto il terzo settore nuove ed altre forme di controllo non condivise e non gestite in modo collaborativo. Che fosse giunto il momento di prendere atto dei cambiamenti intervenuti, semplificare, chiarire e di mettere al pulito il quadro normativo di riferimento era ormai chiaro a tutti e perciò bene ha fatto il Governo a porsi l'obiettivo di avviare un progetto di riforma complessiva di tutto il terzo settore. Un disegno difficile ed ambizioso, un progetto articolato, che presenta molti punti positivi e che, soprattutto, ha tentato di confrontarsi con i cambiamenti avvenuti in questo delicatissimo comparto sociale, culturale è stato accompagnato da un dialogo ed ha aperto speranze ed aspettative, tuttavia, a mio avviso il progetto è tornato a chiudersi in se stesso nella fase finale, nel confronto istituzionale vero e proprio. Si tratta di un vasto disegno di delega e come tale anche pochi cambiamenti possono incidere, poi, moltissimo in fase di svolgimento della delega. Nutro molte buone aspettative, ma il mio giudizio finale non può che essere rimandato alla presentazione dei risultati finali. Nel progetto di riforma è evidente la centralità del tema dell'impresa sociale. Considero questa centralità dell'impresa come una sfida, un modello operativo e di riferimento per gestire servizi complessi, fortemente strutturati ed estesi; ma il modello dell'impresa non può rappresentare un'alternativa obbligata all'associazionismo

generare perdite economiche, tutta la partita delle forme di finanziamento del mondo associativo diviene centrale per la sua continuità e per la sua efficacia operativa. In fondo questo, congiunto alla questione della valorizzazione dell'attività dei volontari, sono due dei nodi fondamentali cui siamo chiamati a rispondere con chiarezza e semplicità; altrimenti facciamo della inutile dialettica su cose astratte che poco hanno a che vedere con la realtà. L'associazione di volontariato deve poter conservare la possibilità di gestire anche servizi complessi avvalendosi anche di specifiche professionalità se organizzati in autonomia, originalmente progettati dalle associazioni o co-progettati con gli enti locali per rispondere a bisogni, sperimentare, innovare il rapporto economico, funzionale e di call con gli enti locali; semplificando

Dice un proverbio che il diavolo si nasconde nelle piccole cose e l'approvazione dell'emendamento al quale mi riferivo: poco più che "una paroletta" ne è l'esempio. Mi spiace anche che tra gli emendamenti approvati in Commissione ce ne sia uno che sopprime il limite di tempo di un anno per la presentazione degli esiti della delega.

non so se sia più avvilente vedere come è stato ridotto questo Parlamento e la democrazia, costretti a legiferare per delega, oppure il fatto che stiamo vedendo il fondo del baratro contro cui fra poco ci schianteremo insieme all'intera Nazione. Queste ridicole e generiche raccomandazioni, che probabilmente il *Premier* neanche leggerà - mi dispiace per il collega Lepri - sono l'ennesimo schiaffo a tutti noi e a milioni di italiani. Abbiamo precedenti eccellenti di come questo Governo abbia consapevolmente ignorato la volontà di questo Parlamento, quando, per esempio, ha inserito nei decreti del *jobs act* la facoltà di licenziamento collettivo che qui, in queste Aule, avevamo chiesto a maggioranza (e votato) di non permettere. Certo non mi stupisco, ma è inevitabile la domanda: a chi giova stare qui a perder tempo? Forse perché siamo solo intrattenimento? Siamo un Parlamento inutile, cari colleghi, una messa in scena o peggio una pantomima. Il copione della seduta prevedrebbe che qua ora si stabilisca di delegare Renzi a riorganizzare il mondo del volontariato e del servizio civile, migliorandolo, bla, bla, bla, bla; ma ecco - arriviamo al punto - la grande idea: trasformare definitivamente il volontariato in lavoro precario e gratuito. Calpestare il valore fondante per un volontario, cioè il gesto disinteressato, riuscendo persino a lucrarci sopra. Sfruttare le persone, mentre costruite la solita piramide di sfruttamento e potere, al cui vertice c'è la "morte nera" delle fondazioni, una superfondazione centrale plenipotenziaria renziana per gestire *in* *toto* contributi pubblici e privati, in modo clientelare (già lo sappiamo), mentre parimenti tagliate sulla spesa sociale, assistenziale e culturale. Non so se è chiaro quali siano i vostri piani, ma non dovrebbe essere difficile capire cosa avete in mente, dal momento che abbiamo visto cosa siete stati in grado di fare con le cooperative, con ricchi appalti gestiti da voi partiti in favore di imprenditori amici e amici di amici, cancellando diritti dei lavoratori e diritti umani in un colpo solo. Abbiamo visto come avete approfittato della possibilità di fare appalti al massimo ribasso, come avete approfittato delle esternalizzazioni, dei lavoratori che vengono pagati 3 euro l'ora dalle vostre cooperative. Abbiamo visto i Buzzi, i Carminati, i volontari-lavoratori o lavoratori-volontari (come volete chiamarli), pagati una miseria con rimborsi in nero, magari *voucher*, mentre i politici corrotti dei vostri partiti si sfondavano di soldi pubblici. Ci ricordiamo la cooperativa La Cascina, i "migranti che fanno fare più soldi della droga", Legacoop e Odevaine, il sottosegretario Castiglione, Non dimentichiamo che queste cooperative svolgono proprio servizi assistenziali e sociali - eh sì! - e che, insieme a tutto il comparto del terzo settore, alle associazioni, alle cooperative sociali e alle ONLUS, oggi sono chiamate a tenere a bada i cittadini bisognosi di servizi (malati, invalidi, anziani, bambini e famiglie), mentre lo Stato li abbandona a se stessi e si demoliscono sanità pubblica, *welfare*, pensioni, scuola, istruzione, ricerca, lavoro, impresa, credito e risparmio. Questo è l'obiettivo: demolire lo Stato sociale e il tessuto economico del Paese, tutto quanto di pubblico e gratuito esiste per i cittadini (e magari anche di efficiente). Si inizia dall'alto, come ha ordinato JP Morgan, quando per le riforme costituzionali vi consigliava di rinunciare a quegli elementi socialisti che impregnano la nostra Costituzione, secondo loro: e perciò riduzione della sovranità del popolo, della possibilità di esprimersi con il voto e con le preferenze, per poi passare al *jobs act* e alla distruzione dei diritti del lavoratori, senza uno straccio di ammortizzatore sociale, complici e conniventi i vostri sindacati confederali, sempre al servizio dei partiti. Con stipendi e pensioni da fame, dopo la legge Fornero, i blocchi alle pensioni, gli aumenti dei prezzi delle bollette, le famiglie italiane, i cittadini giovani e anziani e soprattutto coloro che necessiterebbero di assistenza sono in realtà abbandonati a se stessi. Se in famiglia hai un disabile o un anziano in gravi condizioni di salute,

finanziata da qualche amico di Renzi. Caro cittadino, questi faranno i soldi sulla tua rovina, non hanno alcuna pietà. Lucrare è la loro ricompensa, cioè la ricompensa dei partiti, mentre distruggono il tessuto sociale ed economico per conto e per mandato della *troika*. Quindi? Quindi ricominciamo dall'inizio: bocciamogli il *referendum* costituzionale, riprendiamoci la sovranità, andiamo a votare e poi cambieremo tutto, compresa questa ignobile legge delega, e ridaremo i servizi ai cittadini e la dignità che merita al gesto volontario e disinteressato dei cittadini generosi. generosi. Comprendo che ci sono cose che voi non potete capire, così occupati a gestire attività criminali, così impegnati a fare leggi in favore di banche e speculatori amici e parenti. Per chi di voi non gestisce banche c'è sempre una fondazione pronta. Meno male che vi arrestano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito con attenzione l'evolversi del percorso di riforma del terzo settore e, allo stesso tempo, l'ho seguito con apprensione, dato che la delega va ad interessare un ambito vitale della società, rispetto al quale è vietato sbagliare. Decisivo risulterà l'intervento successivo del Governo, ma innanzitutto determinante sarà l'azione dello stesso Senato nel fissare principi, definire modalità di intervento ed orientare l'assetto e le forme giuridiche ammesse. Vorrei perciò soffermarmi solo su alcuni aspetti critici, che nel testo del disegno di legge non hanno trovato a mio avviso adeguata soluzione e che, se approvati, facilitano l'evolvere di scenari preoccupanti per gran parte dei soggetti del terzo settore italiano operanti nei settori del sociale, del culturale, dell'ambientale, eccetera. Sin dalle definizioni si denota lo scarso rilievo attribuito al profilo partecipativo, in tal modo dichiarando poca attenzione ad un'adeguata *governance* partecipata, democratica e radicata territorialmente. Sottolineo poi la mancanza di sostegno e promozione del testo verso le associazioni ed i soggetti di minori dimensioni, meno strutturati e tuttavia molto radicati territorialmente. Parliamo del 68 per cento di tutti i soggetti censiti censiti dall'ISTAT, che rischiano di vedersi ostacolati e minacciati nella loro stessa esistenza. Nutro ancor più forte perplessità nei confronti di una delle principali novità, novità, l'emendamento governativo che istituisce la Fondazione Italia sociale. In questo caso parliamo di un *unicum* che racchiude in sé finanziatori e risorse da destinare al terzo settore. Innanzitutto, un profilo di criticità mi pare rintracciabile nella natura giuridica di fondazione, la quale, pur avendo una finalità pubblica, avrà natura giuridica privata e quindi non soggetta a determinati obblighi Non condivido nemmeno lo stanziamento iniziale, come hanno già detto alcuni colleghi, a carico dello Stato, di un milione di euro. In barba alle logiche del libero mercato, la fondazione vedrà assicurato fin dalla sua nascita un vantaggio competitivo a scapito degli altri soggetti Non solo: prima si dice alla Nazione che non ci sono risorse, salvo poi tirarle fuori dal salvadanaio per istituire inutili carrozzoni. Tutto questo porta al risultato di calamitare l'area della filantropia, la quale troverà forse troverà forse più consono orientarsi verso un ente preconfezionato strutturato e di respiro nazionale piuttosto che prestare la propria opera di beneficenza a enti di volontariato territoriali. Una logica quindi che allontana il mondo del volontariato dalle caratteristiche ed esigenze specifiche del territorio. Ancor più assurdo è che venga lasciata completa discrezionalità alla fondazione nel determinare le priorità e la scelta dei progetti da realizzare e quindi finanziare. Prima si attraggono risorse su risorse, sottraendole agli attuali soggetti di terzo settore privati, per poi gestirle in modo centralistico penalizzando le iniziative mirate ai territori, e in particolare a quelli svantaggiati. Si tratta di uno schiaffo, a mio avviso al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione, il quale prevede che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»; è il principio che dovrebbe ispirare le istituzioni a creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e ai gruppi sociali l'autonoma iniziativa e l'agire liberamente nello svolgimento della propria attività sociale. In questo senso, meglio sarebbe stato prendere atto della diversa situazione esistente nei territori della penisola e differenziare l'approccio sulla base delle effettive esigenze locali. L'ennesima riforma che volta le spalle ai cittadini dei territori più periferici e svantaggiati, questa volta è ancor più grave in quanto va a colpire l'articolato mondo dell'impegno volontario, ingabbiandolo in un soggetto istituzionale di rango nazionale e quindi, a mio avviso, centralista. Se uccidiamo la volontà di libera iniziativa dei cittadini singoli e associati, se mettiamo a queste realtà i bastoni tra le ruote - o meglio le fondazioni tra le ruote - cosa resterà dell'iniziativa locale? Come dice il presidente Mattarella, è necessario favorire l'opera dei cittadini attivi che in modo libero, autonomo e responsabile contribuiscono a tenere in piedi le istituzioni democratiche, riaffermando la garanzia dell'impegno civico e la libertà associativa quale fattore di crescita della coesione sociale del Paese; parole e concetti condivisibili, ma che difficilmente troveranno terreno fertile a causa dell'imprudente neocentralismo che caratterizza anche l'iniziativa legislativa di cui stiamo trattando. Questa riforma ci restituisce uno scenario deludente, precursore di prospettive non condivisibili e centralista nella sua interezza. Occorre riconoscere nell'azione dei cittadini di organizzarsi volontariamente per dare risposte alle esigenze quotidiane della società la motivazione storica fondativa che ha portato a dare origine a vari soggetti del terzo settore; ma qui non si è stati capaci di cogliere la sfida per gli anni futuri, addirittura arrivando a mettere in discussione l'applicazione del principio di sussidiarietà, dato che non viene assicurata uniformità ed uguaglianza su tutto il territorio. È necessario in tal senso evitare di buttare alle ortiche le esperienze, ad esempio, di lavoro svolto in questi anni dai centri di servizi per volontariato che sono stati punto di riferimento territoriale decisivo. Concludendo, vorrei ricordare al Presidente del Consiglio e al suo Governo che quasi tutte le attività sono svolte da centinaia di migliaia di cittadini che hanno dato un senso alla parola sussidiarietà operando laddove lo Stato è assente o colpevolmente inadeguato. Creare le fondazioni o l'ennesimo poltronificio non farà altro che svilire l'opera di tanti cittadini di buona volontà e di operativa intraprendenza che, per l'ennesima volta, vedranno tradito il loro impegno

Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento, credo che vadano fatte alcune premesse per riuscire a inquadrare il solco entro cui stiamo per legiferare. Nel corso dei secoli il principio di sussidiarietà è stato declinato in due differenti accezioni: accezioni: quella verticale e quella orizzontale. Nella sua dimensione verticale la sussidiarietà è intesa quale principio teso a definire le sfere d'influenza delle singole amministrazioni che operano a livello differente così da fungere quale principale principale criterio ispiratore dell'attività amministrativa. In realtà, nel testo della Costituzione italiana, prima della riforma del 2001, si rinvenivano le tracce del principio di sussidiarietà sia nella formulazione dell'articolo 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale») sia nella lettura sistematica dell'articolo 2 con l'articolo 3, secondo comma («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»). In seno all'Assemblea Costituente, tramite un ordine del giorno del 9 settembre del 1946, Dossetti propose quale principio fondante del nuovo Statuto dell'Italia democratica il riconoscimento della precedenza sostanziale della persona umana intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella. L'ordine del giorno proseguiva affermando che va riconosciuta, ad un tempo, la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità. Pensiamo alla comunità familiare, anzitutto,

È solamente nel 1992, attraverso il Trattato di Maastricht, che il principio di sussidiarietà acquista in modo espresso forza percettiva, comportando comportando naturali riflessi anche per l'ordinamento italiano. Di fatti, l'articolo 3 B del Trattato, nella sua formulazione originaria, prevedeva che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Sulla scorta del principio espresso a livello comunitario anche il legislatore nazionale ha valorizzato in modo esplicito il principio di sussidiarietà verticale, fondando su di esso la garanzia delle autonomie territoriali e interpretandolo come clausola di flessibilità per l'intervento del potere centrale. Una compiuta e definitiva formulazione del principio in questione si ha con la riforma proprio del Titolo V della Parte seconda

«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferiti a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza». Detto comma declina senza incertezze la gerarchia che deve essere seguita al fine di garantire una proporzionata definizione delle sfere di intervento dei vari organi dell'amministrazione. In buona sostanza, il principio affermato è quello in base al quale va sempre preferito il livello di istituzione più vicino al cittadino, in base alla considerazione per cui proprio gli enti più vicini agli interessati sono in grado di soddisfare meglio le loro esigenze. Tuttavia, la mera definizione di un ordine di intervento delle varie amministrazioni statali non poteva essere sufficiente a fornire una risposta efficace alla moltitudine di istanze e bisogni della società che la realtà quotidiana proponeva,

«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». La norma, quindi, delinea perfettamente la diminuzione orizzontale della sussidiarietà, chiamando i cittadini ad attivarsi per lo svolgimento delle attività di interesse generale e gli enti locali, dal canto loro, ad assumere un ruolo di promozione, sostegno e, laddove necessario, sostituzione. La sussidiarietà, con il riconoscimento e la valorizzazione della della responsabilità di tutti i livelli, e cioè sia degli amministratori (sussidiarietà verticale) che della cittadinanza (sussidiarietà orizzontale), crea di fatto un nuovo sistema di gestione del territorio e dei suoi bisogni, modificando profondamente il ruolo affidato ai cittadini. Viene infatti a sorgere una nuova forma di partecipazione alla vita pubblica, che si estende oltre il mero esercizio del diritto di voto e che rende ciascuno partecipe delle sorti della collettività e del bene comune. In buona sostanza, la riforma costituzionale, promuovendo l'azione delle aggregazioni di cittadini e delle associazioni che volontariamente intendono impegnarsi attivamente sul territorio, ammette che l'intervento diretto dello Stato può giungere fino a un determinato livello, oltre il quale è meglio che si lasci l'iniziativa a chi vive direttamente il territorio. Quindi, siamo proprio nello scenario del *welfare mix* o plurale che,

in questo scenario il terzo settore si configura come una modalità positiva e propositiva posta in essere dalla società civile. L'azione società civile. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività. Tali criteri devono caratterizzare anche il terzo settore, che deve pretendere e anche garantire regolamenti chiari per i meccanismi di rappresentanza e partecipazione. Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, in altre parole deve vigilare sull'attività degli enti locali per il rispetto delle procedure, per l'emanazione e l'applicazione di una normativa chiara con regolamenti unici su tutto il territorio nazionale, puntuali e univoci, che non diano adito a interpretazioni diverse nelle varie Regioni. Bisogna necessariamente immaginare dei meccanismi di rappresentanza che siano in grado di dare voce alla diversità di pensiero che esiste nel terzo settore e scardinare i meccanismi negativi di *lobbying* che esistono anche nell'associazionismo.

Signor Presidente, il testo che stiamo prendendo in considerazione e che è stato approvato dalla Camera ormai un anno fa prevede - come tutti sappiamo - una delega in materia di terzo settore, impresa sociale e servizio civile, oltre che una revisione del titolo II del libro I del codice civile sempre in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. Il testo era già stato ampiamente rivisto e modificato in senso - a mio giudizio - migliorativo in occasione del dibattito alla Camera ed è stato ulteriormente modificato positivamente in Commissione.

il terzo settore è un grande patrimonio di persone, di capitale sociale, di fiducia, di interventi: oltre 290.000 associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso (che, tra l'altro, hanno una storia lunga secoli); oltre 4 milioni di volontari e oltre 600.000 dipendenti e lavoratori esterni che arrivano quasi a 300.000. Si tratta di un settore che, secondo le stime dell'ISTAT, dà un apporto di circa 64 miliardi l'anno e, quindi, di un settore importante che si affianca allo Stato e al mercato e, proprio per questo, viene individuato come terzo settore. Il provvedimento in esame interviene su una normativa molto vasta e complessa che si è stratificata nel corso degli anni con molte modifiche, adottate di volta in volta in maniera disarmonica, differenziata, e certamente aveva bisogno

Lo sforzo positivo profuso nei confronti degli elementi di chiarezza che erano necessari è sicuramente apprezzabile. sforzo di semplificazione, di alleggerimento degli aspetti burocratici che coinvolgono tutti questi settori; uno sforzo che in buona parte rinvia ai decreti delegati. su questi, noi richiamiamo l'attenzione di coloro che dovranno dare piena attuazione ai principi, che non sempre sono scritti in maniera chiara e che toccano, con riferimenti molto generici, aspetti molto importanti del terzo settore sui quali avremmo forse voluto una maggiore specificazione. Ho in mente - ad esempio - il fatto che il settore *no profit* in alcuni casi - e lo dico con grande amarezza, ma non possiamo nasconderci questi aspetti - ha ancora

rispettati, neanche da quel mondo che, in realtà, è portatore di valori etici, civili e sociali, che tutti noi apprezziamo ma che, qualche volta, si dimentica di mettere in campo. voglio rapidamente fare riferimento ad alcuni aspetti che - a mio giudizio - sono rimasti ancora non così definiti. Faccio riferimento solo a due aspetti, visto il il tempo piuttosto ristretto che ognuno di noi ha a disposizione. Mi riferisco alla revisione del sistema dei centri di servizi di volontariato, che sappiamo essere un sistema che ha grande ruolo all'interno di questo mondo ma che, probabilmente, poteva essere definito ulteriormente al meglio. In particolare, ricordo uno degli emendamenti sui quali noi contiamo di avere attenzione da parte del relatore e del Governo, che prevede che gli enti del terzo settore, di cui all'articolo 1, comma 1, possano essere coinvolti, non soltanto nella costituzione ma anche nella gestione dei centri di servizi di volontariato. Vorrei, però, dedicare il tempo che mi resta a una delle questioni che mi paiono più rilevanti, nel bene e nel male, che è quella che fa riferimento all'emendamento 9.0.100, del Governo, ovvero l'istituzione della Fondazione Italia sociale.

riconoscere che il Governo ha accolto, riformulando la versione presentata in questi giorni, alcune delle perplessità che, anche in occasione del dibattito in Commissione affari costituzionali, sono emerse, come - ad esempio - il riferimento ai soggetti e ai territori svantaggiati; alla presenza negli organi di governo di un rappresentante del terzo settore; all'introduzione - mi stupisce che chi ha fatto una proposta che vuole essere così innovativa l'abbia trascurata - di sistemi di valutazione e verifica dell'effettivo impatto sociale, che è la frontiera dell'innovazione per tutte le politiche pubbliche e, a maggior ragione, per chi crede di poter avere una grande capacità d'impatto.

soggetti in grado di potenziare la nostra capacità di realizzare interventi innovativi, capaci di avere un elevato impatto sociale e occupazionale. E, quindi, ben venga l'attenzione nei confronti di questo tema. Quello che mi crea ancora dubbi è per quale motivo una fondazione, che viene istituita con l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali,

da mettere a disposizione dei cittadini. Ciò che mi preoccupa, in particolare, è il fatto che mentre, giustamente, si dice che questa fondazione svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico, 9.0.100 si dice che essa può adottare strumenti e modalità di investimento, anche con riferimento alla diffusione di modelli di *welfare* integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico. allora, la frase «rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico?». Non vorrei che ciò aprisse la strada a uno scenario che purtroppo, di fatto, implicitamente già ovvero che l'intervento pubblico si ritrae sempre di più, per varie ragioni, a partire dai problemi della finanza pubblica e, siccome non riesce ad assicurare alcuni servizi, lasciamo la possibilità ad alcune istituzioni private di farlo non solo con fondi privati - cosa che sarebbe assolutamente apprezzabile - ma anche e soprattutto attraverso la raccolta di fondi pubblici. Quindi, si il rischio di favorire il ritiro dell'intervento pubblico, formando un'associazione che poi però si avvarrà di finanziamenti non solo privati, ma anche pubblici.

Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, giunge al nostro esame il disegno di legge per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina L'iniziativa legislativa è stata presa dal Governo, ma in questo caso, a differenza di altre pseudo-riforme, da noi spesso censurate, non si può non rilevare l'utilità e la necessità di siffatta proposta. Infatti, la legislazione vigente in questa materia è notevolmente farraginosa e disorganica, fondandosi la stessa su alcun norme del codice civile e segnatamente su quelle del libro I, titolo II, e su una serie di provvedimenti normativi stratificatisi negli anni. La *ratio* di questo disegno di riforma può quindi ritenersi condivisibile. D'altronde, le materie disciplinate - terzo settore, impresa sociale e servizio civile - sono diventate così strategiche per il nostro Paese, che non era ulteriormente tollerabile il disordine normativo sopra riferito. Solo per ricordare a noi stessi l'importanza del terzo settore, *latu sensu* considerato, basta dare un rapido sguardo ai numeri degli ultimi anni.

Come si vede, si tratta di cifre particolarmente importanti, che meriterebbero approfondimenti e riflessioni ben più ampie di quelle contenute in questa discussione generale. Un'altra riflessione su questi dati può riguardare la distribuzione disomogenea sul territorio nazionale di enti *no profit* e associazioni di volontariato. Quel numero di 681.000 addetti, cui accennavo prima, è ad esempio contenuto per la metà in sole tre Regioni - Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio - così come la maggior parte degli enti si trova nel Nord, poi segue l'Italia centrale, con un Sud che ancora arranca anche da questo punto di vista. Tutte queste considerazioni ci fanno comprendere l'importanza di tale comparto nel nostro sistema economico e sociale. Proprio per queste riflessioni, il nostro compito, ovvero quello di predisporre una delega al Governo per dare una nuova e piena disciplina al terzo settore, è al contempo delicato e strategico. Uno dei principi da confermare, come previsto dall'articolo 118 della Costituzione, recepito nell'articolo 2, primo comma, lettera *a)* del disegno di legge, è certamente quello della sussidiarietà orizzontale. Si pensi - ad esempio - alla forte relazione tra enti locali e soggetti del terzo settore. Nel corso degli ultimi due decenni, il legislatore, confortato dall'avallo dell'opinione pubblica, ha decisamente preferito che taluni interessi generali, siano perseguiti e realizzati da enti o formazioni sociali presenti sul territorio, piuttosto che dalle amministrazioni pubbliche. Una coerente applicazione di siffatto obiettivo è stata, in tal senso, la legge n. 328 del 2000, con la quale si è riformato il sistema dei servizi sociali, da molti colleghi menzionato. Come si sarebbero potuti realizzare gli ambiti territoriali dei servizi sociali con le sole energie umane e finanziarie dei singoli Comuni associati o delle aziende sanitarie locali? È questa la domanda che ci possiamo porre a proposito della legge n. e soprattutto dal 2011 in poi, quando i tagli nei confronti degli enti locali e dei Comuni sono stati così forti che per i piccoli Comuni è stato proprio difficile pensare ad un *welfare* locale.

Oggi faticosamente i cosiddetti piani d'ambito iniziano a dare qualche risposta solo grazie all'apporto dei soggetti cui è indirizzato il presente disegno di legge, a fronte dell'impossibilità dei Comuni di poter realizzare un proprio servizio di assistenza sociale.

Cosa sarebbe successo in quel settore senza l'apporto dei volontari? Proprio qualche giorno fa in Aula ho ricordato il ruolo decisivo del volontariato, insieme alle Forze armate e di polizia, per fronteggiare il complicatissimo problema dell'accoglienza umanitaria e sociale di tutti quei diseredati sbarcati nel corso degli ultimi venticinque anni. Se la risposta a siffatto problema fosse stata quella delle amministrazioni pubbliche, l'Italia si sarebbe contraddistinta in negativo, ben peggio di quanto stia facendo la Grecia a Idomeni (per usare un esempio abusatissimo delle ultime settimane). E potremmo continuare citando l'importanza del terzo settore nella soluzione delle varie emergenze di protezione civile, purtroppo sempre frequenti nel nostro Paese; anche in il terzo settore diventa, in certi momenti, non sussidiario, ma sostituivo della risposta pubblica. Analogamente occorre riflettere sul ruolo delle fondazioni bancarie, interlocutrici necessarie del Governo centrale, come delle università e degli enti locali. L'importanza di tali associazioni, imprese e fondazioni ha condotto alla condivisa opinione della necessità di una riforma e attualizzazione del sistema di norme finora disordinatamente emanate dal legislatore, come dicevo all'inizio. Molti dei principi e dei criteri di delega rinvenibili nel testo al nostro esame vanno nella direzione giusta. Non si può non rilevare, però, in questa sede, l'eccessiva ampiezza della delega stessa. Ma questo è un difetto che molte altre volte abbiamo dovuto evidenziare, sia perché il Governo spesso ricorre a leggi delega, sia perché

quanto importante sia questa legge, per via dell'incertezza sull'*iter* degli emendamenti che l'ottimo relatore Lepri ha predisposto nelle ultime ore e dei consequenziali subemendamenti. Attendiamo, quindi, lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea per dare un giudizio più compiuto su alcune questioni ancora non definite, così come già evidenziato nei lavori preparatori, specie per quanto attiene al ruolo e alle funzioni della Fondazione Italia sociale,

Oggi discutiamo l'ennesimo disegno di legge di iniziativa governativa, che presenta sempre lo stesso identico schema e purtroppo caratterizza molti dei provvedimenti dell'Esecutivo: accentrare sempre di più il potere legislativo verso lo Stato, depotenziando le competenze e le funzioni delle Regioni e degli enti locali; ma soprattutto mettere in moto quel processo di cassa di risonanza mediatica di cui Renzi è il campione *superstar*, presentando come riforma ciò che in sostanza si rivela un puro esercizio di stile. Prima di ogni altra argomentazione è doveroso criticare la *ratio* stessa del presente disegno di legge, che intende classificare come terzo settore tutto ciò che non fa parte dei primi due. I principi generali del provvedimento, infatti, delineano un sistema del *no profit* sostitutivo del settore pubblico e alimentato da agevolazioni fiscali e donazioni dei privati. È la prospettiva del *welfare* residuale, in cui l'impresa sociale potrà intervenire anche in settori quali la formazione universitaria e l'assistenza sanitaria. In sostanza, si apriranno ancora di più le porte alla privatizzazione dello Stato sociale, e in particolare in due settori che sino a oggi hanno comunque mantenuto un forte impianto pubblico: la sanità e l'istruzione. La rilevanza assunta negli ultimi anni dal terzo settore per l'economia e la società italiane è nota ed è stata dimostrata anche dai risultati del censimento ISTAT sulle istituzioni *no profit*: rilevanti, appunto, sono le risorse umane impegnate nel settore,

Infatti, rispetto al 2001, è raddoppiato il numero di istituzioni e collaboratori esterni, con un incremento del numero dei collaboratori. Si parla di quasi 80 miliardi di euro di entrate, corrispondenti al 3 per cento del PIL nazionale. Si mascherano sotto l'etichetta del *no profit*, purtroppo, anche organizzazioni molto simili a imprese private, che approfittano dei benefici fiscali. fiscali. Intervenire per rafforzare il terzo settore in un momento storico come questo, in cui inchieste giudiziarie come quella di Mafia Capitale hanno fatto emergere con chiarezza una commistione tra politici corrotti, cooperative sociali e associazioni criminali, senza prevedere formule di contrasto a queste devianze del settore, appare a noi totalmente irragionevole. Il presente disegno di legge prevede soluzioni inadeguate, come quella di accentrare le competenze a livello statale istituendo il registro unico, coinvolgendo l'Agenzia delle entrate nell'azione di controllo sull'andamento delle attività, e soluzioni di portata relativa, come l'aumento del tetto massimo per le detrazioni fiscali sulle donazioni ad Onlus o interventi disomogenei rispetto al contesto della riforma, come la trasformazione del servizio civile in servizio civile universale, senza che sia dichiarato cosa in realtà si intenda e che cosa sottostà a tale servizio civile universale. Le disposizioni nell'ambito del servizio civile appaiono infatti sganciate dal contesto del disegno di legge delega e non organiche. Se il Governo ipotizza di esercitare questa delega in bianco, per normare la partecipazione degli extracomunitari a questa attività, vìola palesemente il rispetto della sovranità nazionale e il concetto stesso che devono invece caratterizzare un istituto come quello del servizio civile, nato dalla volontà di istituire un sistema alternativo alla leva obbligatoria. Vedete colleghi, la previsione di un registro unico del terzo settore al fine di favorire la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale è in contrasto con il rispetto delle prerogative delle Regioni, ai sensi anche della disciplina costituzionale prevista dal Titolo V. Ci saremmo aspettati una riforma del terzo settore in grado

non hanno bisogno del registro unico del terzo settore, ma piuttosto di essere aiutate, perché la burocrazia che purtroppo devono affrontare è sempre maggiore.

Nella definizione si parla di realizzazione e sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di terzo settore: praticamente il classico carrozzone all'italiana.

Abbiamo visto, purtroppo, nella nostra triste realtà, come dietro alla collaborazione, al volere aiutare gli altri, ci sia semplicemente un voler approfittare

agli studenti e ai docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Michele dell'Aquila» di San Ferdinando di Puglia, della provincia di Barletta-Andria-Trani. *(Applausi).* È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Signor Presidente, bisogna riconoscere al Governo e alla maggioranza di essere un vero ufficio complicazioni affari semplici. Il Governo, ormai due anni fa, presenta un disegno di legge delega sul terzo settore con l'immancabile annuncio: «Esiste un'Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone. È l'Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo *no profìt*, delle fondazioni e delle imprese sociali. Lo chiamano terzo settore, ma in realtà è il primo». Questo è l'annuncio roboante. Molti di noi che abbiamo dedicato una buona parte della vita al mondo dell'associazionismo abbiamo tuttavia ben sperato, tuttavia ben sperato, anche perché l'*iter* parlamentare è iniziato alla Camera dei deputati dove sono presenti illustri esponenti proprio di quel mondo, presidenti di grandi associazioni, una presenza mai vista, un grande riconoscimento politico. Dunque, ci saremmo aspettati finalmente una legge quadro sul terzo settore che potesse mettere insieme le diverse discipline e rafforzarne il ruolo. È sempre stato complicato il rapporto tra terzo settore e normativa. Per anni si è fatto riferimento al codice civile e a tante altre norme per lo più fiscali, per interpretazione estensiva. Nel 1997 viene approvato il decreto fiscale n. 460 del ministro Visco: una pietra miliare, finalmente un primo passo dove si stabilivano importanti criteri fiscali per il riconoscimento di agevolazioni identificative e si individuavano criteri per definire le varie tipologie di *no profit*, e uno su tutti: la partecipazione dei cittadini, il ruolo dei soci.

di un coarcevo di norme che avrebbe avuto necessità di armonizzazione e di una lettura aggiornata alla luce di cosa è realmente questo settore. Oggi il vasto e ricco mondo dell'associazionismo diffuso, del volontariato e del *no profit* è un pezzo importante non solo della nostra economia - com'è stato più volte detto - ma sopratutto del nostro tessuto democratico, che ha antiche e solide radici nel solidarismo e nella mutualità italiana. Nella seconda metà dell'800, a seguito delle grandi e profonde modificazioni economiche e sociali legate all'industrializzazione e alla formazione dello Stato unitario, si sviluppa il movimento associativo delle classi lavoratrici. Nascono le prime società di mutuo soccorso (SMS) e le società operaie di mutuo soccorso, che si occupano di assistenza, beneficenza e mutualità, diventando un punto di riferimento per la nascente classe operaia. operaia. Influenzate da ideali mazziniani, anarchici e socialisti, le SMS perdono rapidamente la apoliticità delle origini, anche se, in assenza di una linea politica comune, alcune si dedicano esclusivamente alla beneficenza e al mutuo soccorso, mentre altre scelgono di impegnarsi attivamente a fianco dei lavoratori nella loro battaglia contro lo sfruttamento. In nome della mutualità, della giustizia e della libertà, le SMS diventano soggetti essenziali per la creazione di luoghi di ritrovo, di cultura, di istruzione e di formazione politica, favorendo nell'allora nascente proletariato la presa di coscienza della propria condizione, sia politica che sociale. I corsi di istruzione e di alfabetizzazione degli operai trovano piena organizzazione nelle società di mutuo soccorso. Sono palestre di democrazia, luoghi di ritrovo, istruzione e cultura. Nel corso degli anni, il fascismo con le leggi repressive, la lotta di liberazione e la nostra Costituzione segnano tappe importanti per la trasformazione dell'associazionismo laico e cattolico, attraversato da grandi fermenti sociali che sa interpretare, rappresentare e a volte anticipare. Il radicamento territoriale e sociale è la sua principale forza, pur con le specificità regionali; una rete diffusa di spazi aperti dove i cittadini si incontrano, condividono interessi e passioni, fanno attività nell'interesse della comunità, promuovono la partecipazione alla vita pubblica. Oggi, quando parliamo di terzo settore, siamo dinanzi a un pullulare di esperienze associative e cooperative, che in questi anni hanno contribuito a costruire un pezzo importante del nostro *welfare* sociale, culturale e ricreativo. Tutto questo è accaduto in piena collaborazione con gli enti locali e le Regioni, sperimentando forme nuove di intervento pubblico, ma senza mai tradire il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione; quel principio in base al quale alcune funzioni pubbliche attività di interesse generale possono essere svolte da organizzazioni più vicine ai cittadini, ovviamente nel pieno rispetto dei ruoli e dei poteri diversi; i poteri di indirizzo, programmazione e controllo sono tutti pubblici, senza mai sostituirsi. Quando parliamo di attività e funzioni pubbliche, parliamo oggi di corsi di italiano per stranieri nelle scuole (il famoso L2), attività culturali, spazi gioco, asili nido, centri di prima accoglienza, sportelli legali informativi, doposcuola per ragazzi, cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari, interventi di solidarietà sanitaria, raccolta fondi, corsi sportivi, di musica, ballo, cultura e di enogastronomia, corsi di economia sociale, corsi di educazione sessuale nelle scuole, tutela e prevenzione ambientale, prevenzione sanitaria: insomma, un elenco infinito. Si tratta di attività realizzate da grandi, medie e piccole cooperative, associazioni di volontariato e promozione sociale, da Onlus: un fitto bosco di esperienze e di sperimentazione che non poco ha contribuito a costruire lo Stato sociale italiano, a costruire cittadinanza, battaglia per i diritti. Ogni esperienza è una ricchezza di pratiche, studi, di lavori ai quali in molti casi è stata totalmente delegata la sperimentazione e l'innovazione sociale degli enti locali, al punto che oggi possiamo riconoscere senza alcun dubbio l'utilità sociale pubblica per quei "circolini" che spesso sono l'unico presidio sociale in tanti piccoli centri, in frazioni dove la sera spesso non è aperto nessun altro luogo di ritrovo. Quel circolo svolge un ruolo importante e nessuna attività di profitto, anche quando l'unica attività spesso è quella di essere un bar o un piccolo spaccio. un mondo grande, una ricchezza incredibile, una grande umanità e tanta generosità che avrebbe dovuto trovare piena valorizzazione nel disegno di legge in esame. Per questo è inaccettabile che non si sia utilizzata detta occasione per sciogliere quei nodi che avrebbero aiutato a fare chiarezza, a dare regole certe su quali - ad esempio - sono le attività istituzionali e quelle connesse, per riconoscere le giuste agevolazioni anche fiscali; dire con chiarezza che le attività dove c'è corresponsione di denaro sono funzionali alle attività istituzionali e non al profitto. un errore parlare di attività d'impresa non prevalente, perché automaticamente riconduce all'idea di furbizia e di evasione, e lo abbiamo sentito in quest'Aula. Non c'è alcuna valorizzazione e non c'è riconoscimento del valore sociale delle attività istituzionali e persino del valore sociale indiretto di quelle commerciali. una terminologia che porta a dubbia interpretazione quando, all'articolo 6, si parla di impresa sociale e la destinazione degli utili deve essere prioritariamente destinata allo svolgimento delle attività statutarie. Dunque una parte non prioritaria degli utili può essere ripartita? E si rinvia ai decreti attuativi l'individuazione dei settori di impresa, cosa che sarebbe stata urgente da fare. L'impostazione del disegno di legge è tutta economicista economicista (si riprende il criterio di economicità, si parla di iniziativa economica privata) e anche molto giustificazionista, dimenticando di dare cittadinanza e valorizzazione alla partecipazione dei cittadini, alla partecipazione attiva di tutti coloro che scelgono di mettersi insieme per progetti di utilità sociale, per un'idea di condivisa socialità, cultura, impegno civile: criterio fondamentale per spiegare il senso e la natura giuridica del terzo settore. Partecipazione e autorganizzazione sono concetti che il testo in esame fatica a riconoscere pienamente, se non in senso rivendicativo e di controllo di trasparenza e correttezza, avallando il luogo più che comune che il terzo settore è un po' come Mafia Capitale. La cooperazione ha solidi valori e non è tutto malaffare e ruberie. Tutto questo è frutto di non conoscenza, di populismi e di semplificazioni. Tuttavia, nemmeno si può pensare che una qualsiasi impresa che fa investimenti nel sociale sia da definirsi come un'impresa sociale. È un errore.

non ha risorse per pagare campagne elettorali o la politica; è fatto di cittadini che donano, di cammini collettivi. Certo, deve essere una battaglia comune quella contro le truffe, le false cooperative, le false associazioni, ma la trasparenza degli atti, dei bilanci, dei rendiconti e dei progetti è una richiesta forte che viene da quel mondo e non è considerata in modo punitivo. E non è una novità, perché molte di quelle norme sono già in vigore dal 1997. Non si capisce, invece, perché non c'è stato nessun impegno per un contratto tipico di settore. Troppe diverse sono le tipologie contrattuali, diverse le retribuzioni; troppo precariato. Per un settore che viene considerato il primo settore economico non è accettabile non aver posto tra le priorità i lavoratori, il lavoro e la sua qualità. Da tempo viene chiesto di riconoscere il valore del volontariato tutto, eliminando vetuste classificazioni legate ai luoghi associativi dove si svolge e alle classificazioni legislative ingiustamente punitive, distinguendo tra gratuità e volontariato. Il volontariato, in qualunque modello *no profit* si realizza, ha tutto lo stesso alto valore etico, sociale e di impegno umanitario. Per intenderci, è volontariato quello di chi va a distribuire i pasti alla mensa popolare, così come è volontariato quello di chi organizza la stessa mensa ma in un'associazione di promozione sociale. In questi giorni, dinanzi alla tragedia umanitaria che assistiamo ai confini greci, alcune grandi associazioni si stanno mobilitando per raccogliere materiali e beni di prima necessità e soccorso, una forma di grande volontariato collettivo. Ancora una volta, però le idee sono confuse e gli annunci sempre meno delle aspettative. Tutto diventa più nebuloso quando improvvisamente il Governo ha presentato pochi giorni fa in Commissione e venerdì in Aula la proposta della Fondazione Italia sociale, un'operazione di filantropia umanitaria con l'intento di utilizzare finanziamenti pubblici,

furtivamente in Commissione, e poi c'è stato l'emendamento ritirato. Non c'è stata nemmeno l'opportunità di chiarirci i dubbi che sono nati dinanzi a questo strano emendamento.

ma chiarisce bene che l'intento del Governo non è il riconoscimento sociale, etico e culturale dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, ma è fare una grande operazione di *fund raising* tra i colossi della finanza, dell'industria. nulla di male, ma non era questo il testo per discutere di una fondazione Paese per drenare risorse dai privati a fini umanitari. Ci chiediamo perché questa proposta non sia stata presentata in un disegno altro che prevede la creazione di una fondazione pubblica, uno delle tante. Forse è solo una conferma che in questa discussione ci sono due livelli: quello parlamentare, che ha cercato, nostro malgrado, di coinvolgere i soggetti protagonisti, pur con visioni differenti, e quello del Governo, che invece evidentemente pensa ad un'operazione di grande solidarietà, ma che è altro. Si dimentica che oggi il terzo settore settore è fatto dalla libera scelta di donne e uomini che si mettono in gioco per un percorso collettivo di autogestione e di emancipazione, pur nelle forme simil-societarie oggi nascenti. Sono cittadini che condividono idee positive di cultura, solidarietà, impegno civile, pace e giustizia sociale e diritti umani. Insieme costruiscono un'altra idea di società e contribuiscono nei fatti a cambiarla. La vostra impostazione, invece, risente di un forte retaggio culturale antico. Nel mondo si sviluppano forme di volontariato e condivisione di progetti addirittura in forma collaborativa via *web* (pensate al *crowdfunding* o allo sviluppo di piattaforme *software web* fatte

civica. Non fa semplicemente carità. E questa è la profonda differenza culturale che non riuscite a cogliere all'interno di questo testo.

sono riferite al principio di sussidiarietà che abbiamo voluto elevare a rango costituzionale

dalle molteplici attività che entro quella definizione sono comprese e che vorremmo rendere quanto più efficienti, trasparenti

Tuttavia, a coloro che sottolineano le pur ricorrenti patologie che si sono manifestate in questo ambito, vorrei ricordare

ciò che ricaviamo dalla nostra storia, cioè da quella legislazione dei primi Governi dello Stato unitario con cui si volle pubblicizzare molte opere pie. Non ne derivò

nel complesso sottraemmo a quelle opere pie quel calore relazionale che dà loro un vantaggio competitivo rispetto

si dipanò in questi enti è lì a dimostrare la non scontata efficienza della gestione pubblica rispetto alla cosiddetta gestione privato-sociale.

è compiuta l'integrazione territoriale tra servizi sanitari, servizi sociali e servizi assistenziali. Questa integrazione si realizza perché la relativa spesa viene riunita nelle aziende territoriali. Gli stessi enti locali conferiscono la spesa socio‑sanitaria e assistenziale alle aziende sanitarie territoriali con contabilità separata direttamente da essi vigilata, ma tale da integrarsi compiutamente con la spesa sanitaria e sviluppare

Le vie dell'efficienza chiedono libertà e responsabilità, anzi - aggiungo - libertà, responsabilità e trasparenza. Mi riferisco in particolare all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, laddove una regolazione invasiva, richiamando il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, vorrebbe porre un tetto del 20 per cento superiore ai minimi salariali dei contratti collettivi di riferimento per quanto riguarda i dipendenti di questi enti. Credo che in questo modo non si consentirebbe agli enti stessi di reperire sul mercato quei medici, infermieri, informatici, biologi, esperti di contabilità e bilancio e così via che appaiono più confacenti a perseguire lo scopo sociale. Dobbiamo lasciare libertà contrattuale, altrimenti violeremmo un principio di pari trattamento per quei lavoratori che appartengono sempre al settore privato; dobbiamo cercare di garantire principi di trasparenza, di proporzionalità e nel complesso il contenimento dei costi fissi, di quei costi di supporto

modificare l'articolo 4, lettera *e)*, con principi di delega di carattere più generale, non certo riferentisi a quel decreto legislativo 4 dicembre n. 460, 1997, peraltro rivelatosi inefficace. Concludo con un riferimento al testo, laddove, a proposito degli appalti pubblici, impone che non si adottino criteri peggiorativi per i lavoratori rispetto ai contratti collettivi. Se questo significa la cosiddetta clausola sociale, ricordo che, recentemente, tanto l'Autorità anticorruzione quanto l'Antitrust hanno spiegato l'incostituzionalità della cosiddetta clausola sociale, perché essa non può impedire il perseguimento di obiettivi di efficacia e di efficienza; cioè vale fino a che non vi sia un'offerta migliore dal punto di vista dell'organizzazione di quel servizio, tale da essere di maggior vantaggio per il perseguimento del bene comune.

quando parliamo di volontariato ci riferiamo a una grandissima ricchezza presente in Italia, perché quei numeri ci parlano di quante persone tolgono qualcosa a loro stessi, alle loro famiglie, al lavoro o al tempo libero per dedicarsi ad altri.

Potrei citare tantissime esperienze sociali del primo volontariato, quindi di volontariato vero, puro, bellissimo, presente in molte città italiane,

parola sussidiarietà. Noi sappiamo che quando si parla di ciò si fa riferimento ad una doppia sussidiarietà. La sussidiarietà verticale, che vuol dire Stato, Regioni, Comuni, e la sussidiarietà orizzontale, che è quella che porta i Comuni, le istituzioni più vicine ai cittadini,

Ma non c'è niente di più centralista di quella fondazione; non c'è niente che vada più contro il concetto di sussidiarietà di cui parlavamo prima e, ancora prima del concetto di sussidiarietà, inserito nella Costituzione, contro il concetto di generosità,

Poiché rappresentiamo forze politiche che amministrano il nostro Paese, mi chiedo come non vi sia venuto in mente di chiamare, non solo le associazioni più piccole delle città per sentire le loro esperienze, ma di costruire questa riforma insieme? Il volontariato è di tutti.

della povertà, dell'inclusione sociale. Ma il volontariato è anche lo sport e tanto altro ancora. Ma voi avete mai parlato con un genitore preoccupato perché ha il figlio diversamente abile? Quelle sono le associazioni che bisogna ascoltare. Io voglio sapere lì cosa si fa, come si applica lì il concetto di sussidiarietà. Mi rivolgo al Sottosegretario perché, anche se naturalmente è più importante che parli al telefono, dimostra come noi dobbiamo dire di no alla delega in bianco al Governo, perché è disinteressato a tutto. Credo che non sia un bell'esempio, non perché parlo io, ma perché lo fa quando parlano tutti. Chiedo al Parlamento se va bene così,

caso parliamo veramente di tanto volontariato che si fa nelle città, di tante cose che le amministrazioni comunali, anche per i tagli e per la scarsità delle risorse, non riescono più a fare. a fare. Poiché non si riesce più a farle e il Governo vuole creare anche la fondazione centralista, chi le farà, quando non verranno più fatte dalle persone che lavorano in queste associazioni?

tutti noi conosciamo l'importanza del terzo settore e di tutto l'insieme delle attività che si caratterizzano per essere *no profit*. Tale settore nel corso del tempo ha acquisito un ruolo di fondamentale importanza nella società moderna e riveste oggi un peso economico notevole nel nostro Paese. Come

Soprattutto dopo la terribile crisi economica che ha colpito l'Europa e il resto del mondo, anche a causa degli scenari di guerra presenti, dove i poveri sono sempre più poveri, il problema dei migranti si aggrava ogni giorno e il malcontento sociale continua a diffondersi, ecco che il terzo settore rappresenta una possibile risposta alle sofferenze e ai malesseri dei cittadini. In molti casi a porre un freno a tali angosce e a problemi di varia natura e specie, che colpiscono in particolare i cittadini più svantaggiati, vi è stata la forza del volontariato, delle associazioni, delle imprese sociali, delle società di mutuo soccorso e delle cooperative, che hanno fatto molto in questi anni e continueranno a farlo anche nel futuro. In questo quadro si inserisce il provvedimento oggi all'ordine del giorno, che è il risultato di un lungo percorso di elaborazione ed analisi, iniziato nel maggio del 2014, con una consultazione pubblica

la riforma sono la spinta verso la trasparenza, la rendicontazione, la qualità della *governance* e la valutazione d'impatto. Più in particolare, l'obiettivo del provvedimento è, da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata. Tutto questo, allo scopo di valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno. Dall'altro lato, invece, c'è l'obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina della materia, caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile. ciò per permettere ai singoli soggetti coinvolti di non rimanere imbrigliati e frenati da ostacoli burocratici che ne impediscono la loro essenziale attività sociale. Durante l'esame in Commissione affari costituzionali del Senato, con il poderoso lavoro del relatore Lepri, che ringrazio, sono state inserite importanti novità rispetto al testo approvato alla Camera. Ad esempio, nell'articolo 1, la definizione di terzo settore è stata resa più completa, in modo da ricomprendere in essa tutte le varie componenti e anime di questo mondo. La nuova formulazione prevede che: «Per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Non solo vengono specificate le finalità ma anche le attività quando si prevede che esse «promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi». Per quanto riguarda il tema del lavoro, segnalo che durante l'esame in Commissione sono state effettuate alcune importanti ed opportune modifiche: mi riferisco agli obblighi di trasparenza e informazione, che sono riferiti non solo agli associati ma anche ai lavoratori. Ritengo inoltre di grande importanza la previsione inserita inerente la garanzia che negli appalti pubblici le condizioni

Senza dimenticarci delle norme inserite per la revisione del servizio civile universale, che rappresenta una fabbrica di capitale sociale, una palestra della cooperazione, che oggi manca nel nostro Paese. In questo senso, è importante l'apertura del servizio, prevista in Senato, agli stranieri regolarmente soggiornanti che, come ricordato dal relatore Lepri, risolve il problema posto da alcune sentenze su questo tema. Detto questo, se, come ricordato, tra le finalità vi è quella di creare un unico quadro normativo del settore, è nel provvedimento una opportunità più grande da cogliere: far diventare il terzo settore, il primo settore del nostro Paese, come affermato dal nostro Presidente del Consiglio. perché esso mette al centro la società; perché consente e migliora la coesione tra gli individui e il benessere dei cittadini; perché la politica ne è strumento, per la sua crescita e il suo sviluppo. Con questa chiave di lettura, possiamo dare una visione innovativa della realtà che ci circonda, diversa da quella attuale. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo infatti pensato che l'interesse generale, il bene comune, l'interesse pubblico fossero solamente un affare riservato alle amministrazioni pubbliche e da loro dovesse essere gestito. Ma non è così. Tali questioni, che riguardano i cittadini, devono essere gestite anche dai singoli stessi che si organizzano, tra di loro, in diverse forme e modi, e si dedicano ad attività di interesse generale per finalità pubbliche, imprenditoriali o solidaristiche. Per questo la riforma in corso ha come idea alla base l'abbattimento delle barriere tra mondo delle istituzioni, mondo del terzo settore e mondo delle imprese. L'ente pubblico oggi, o non ha o non ha le possibilità economiche, o non ha le informazioni per conoscere i bisogni della società civile, e spesso la burocrazia degli uffici non capisce il territorio. Parimenti, il mondo dell'imprenditoria ha le risorse, ma spesso manca di una strategia comune di intervento. Infine, vi è la società civile, che sa come evitare il paternalismo assistenzialistico, ma manca di uno *status* giuridico riconosciuto, sulla cui base agire. È necessario che questi tre mondi interagiscano tra di loro e ciò può essere possibile grazie alla sussidiarietà circolare. È questo il principio organizzativo cui si deve ispirare il *welfare* civile del futuro. Fin qui sulla base dell'articolo 118 della nostra Costituzione, abbiamo declinato la già ricordata sussidiarietà come verticale (decentramento amministrativo) o come orizzontale (*welfare* plurale, nelle mani dell'ente pubblico, spesso costretto ad adeguarsi al regime di massimo ribasso). La sussidiarietà circolare permette invece, come si è detto, l'interazione sistematica dei soggetti: sulla base di protocolli stabiliti per definire le priorità di intervento, essa connette il settore pubblico e quello imprenditoriale con la società civile, consentendo di trovare le modalità di gestione più efficaci per raggiungere obiettivi condivisi. Non si tratta di una utopia. Questa riforma è il primo passo verso questo nuovo sistema. Essa si inserisce in un disegno più grande, che si accompagna alla riforma del lavoro e della pubblica amministrazione. Il Governo Renzi e il PD hanno in questo senso cambiato verso: hanno ribaltato la prospettiva del rigore e della politica troppo attenta alle logiche dello *spread* e del debito pubblico e ben poco al *welfare* civile, facendola uscire dai Palazzi per ricollegarla alla società e alla comunità degli individui. non è stato fatto solo questo; si fa per dire e vorrei rassicurare il collega Airola: sono state anche reinvestite le risorse economiche sulle voci sociali dopo anni di tagli. Penso alle risorse per il Fondo sociale, sul servizio civile, sul 5 per mille, sulla buona scuola, sul dopo di noi, sulla cultura e sul provvedimento che prevede una misura strutturale contro la povertà, all'esame alla Camera. Infine, penso ai provvedimenti sulle donne. donne. Le cito non a caso, perché sono le donne ad essere direttamente interessate a questo provvedimento. Sono loro a mettere più impegno nel sociale. Esse dedicano una media di 18,5 ore settimanali a tale attività, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT. Per loro il volontariato e l'attività sociale rivestono un ruolo importante, anzitutto perché si tratta di un ambito in cui è possibile rompere determinati steccati culturali e ideologici, e poi perché le donne vedono nel terzo settore anche possibili risvolti professionali. Concludo, signor Presidente e colleghi: per i motivi esposti e per il contenuto delle norme in esame, credo che la sfida messa in campo oggi con questo provvedimento sia ambiziosa e sicuramente sarà importante il successivo esame dei decreti attuativi, che entreranno nel vivo della materia e ne declineranno il successo. Non bisogna però dimenticare che, a prescindere dalle norme e dalle disposizioni descritte, questa riforma sarebbe poca cosa senza gli attori che ne fanno parte. Questa istituzione oggi, con l'esame di questo provvedimento, ha l'occasione di esprimere tutto il suo riconoscimento nei confronti delle migliaia delle migliaia di addetti e dei milioni di volontari che ogni giorno, con fatica e dedizione, svolgono il loro lavoro nel settore del sociale, con il massimo dell'impegno e della loro professionalità. Detto ciò, ritengo quindi che con l'approvazione di questa norma, vi siano tutte le premesse per conseguire un obiettivo di ampia portata per riformare un settore che da troppo tempo attendeva e richiedeva un intervento organico, così strutturato.

nell'impulso che si vuole dare a tutto il mondo associativo e volontario, e in particolare all'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, ultimo comma, secondo cui le istituzioni della Repubblica favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà. Dunque, il riordino e la revisione sono guidati da questo principio essenziale, che è rimasto in gran parte contenuto sicuramente nella Carta costituzionale riformata nel 2001, ma che non ha trovato poi piena attuazione nelle norme successive. La seconda sottolineatura riguarda l'introduzione del registro unico, su cui diversi interventi Oggi abbiamo una moltiplicazione dei registri che non consente né al cittadino singolo né alle istituzioni pubbliche di avere un'esatta contezza di cosa sia questo mondo. In questa non chiara identificazione, e quindi opacità, si possono nascondere anche quei fenomeni distorsivi che diversi interventi hanno evidenziato. Dunque, il registro unico sarà il modo per rendere trasparente, per il cittadino singolo e per le istituzioni, chi sono questi soggetti, che cosa fanno, chi li guida e come operano in un principio di totale Non sarà obbligatorio iscriversi a tale registro; ci si iscriverà se si vorrà godere di alcune norme di vantaggio che già le leggi esistenti e questo disegno di legge prevedono. Terzo punto: la delega contiene la delega contiene una norma di revisione della legge sul servizio civile. È un punto particolarmente qualificante, in quanto si vuole fare un investimento sui giovani in servizio civile che nel medio-lungo periodo porterà linfa nuova, generazioni nuove proprio nel campo associativo, volontario, cooperativo e mutualistico. Sullo sfondo c'è anche la proposta, recentemente lanciata dal Governo, di arrivare ad un servizio civile europeo. Un quarto punto è la revisione delle norme sulle imprese sociali. Si vuole facilitare, sostenere, una nuova imprenditoria sociale che si accompagna a quella esistente, prevalentemente di natura cooperativa, in grado di affrontare, con una finalità sociale, risposte ai tanti bisogni che oggi non trovano una risposta appropriata. Infine, sul tema delle risorse, vorrei sottolineare che tra la legge di stabilità del 2015, quella del 2016 e

stabilizzato il 5 per mille per un valore di 500 milioni, che è destinato proprio a gran parte di queste realtà associative e volontarie. Nel luglio istituito, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di garanzia rotativo per sostenere gli investimenti delle cooperative e delle imprese sociali. Nella legge di stabilità ci sono quest'anno, per la piena applicazione di questa riforma, 140 milioni; nei prossimi anni 2017 e 2018 sono È stato inserito, proprio nel testo all'esame dell'Assemblea, un fondo per lo sviluppo dei progetti delle realtà associative e volontarie per un valore di 17 milioni. Infine, nella legge di stabilità per il 2015, è stata accresciuta la soglia sulla quale può essere esercitata una detrazione fiscale per le erogazioni liberali, passando da 2.065 euro a 30.000 euro. Si tratta quindi di revisioni normative, di innovazioni normative e di impulso attraverso risorse per far sì che quella norma costituzionale, secondo cui le istituzioni hanno programmaticamente il compito di favorire lo sviluppo, la nascita e la piena realizzazione di questa capacità dei cittadini, singoli ed associati, di perseguire attività di interesse generale, possa trovare un pieno compimento. Si tratta dunque di una norma che richiederà certamente decreti legislativi ed applicativi, che il Governo intende emanare nel più breve tempo possibile e sicuramente entro i termini stabiliti dalla norma che andiamo adesso a votare.

al quale si riferiscono. Pertanto, non sono ammissibili emendamenti volti a sostituire integralmente il contenuto dell'emendamento principale trasformandone l'oggetto e la portata precettiva al punto di costituire un emendamento alternativo rispetto a quello principale. Inoltre, conformemente alla prassi costante in materia di emendamenti, risultano inammissibili le proposte presentate *ioci causa*, quali le indicazioni di specifici toponimi. Per tali ragioni, la Presidenza dichiara inammissibili i subemendamenti da 1.210/1 a 1.210/6,

da 9.0.100/1 a 9.0.100/3, nonché da 9.0.100/8

nella definizione di un terzo settore volto alla produzione sociale, cioè di beni, servizi e mutualità senza fine di lucro, le imprese. imprese. Ancorché intervengano in ambito sociale, queste sono attività economiche che hanno la finalità di produrre una ricchezza per l'imprenditoria. Noi riteniamo che non si possa fare lucro. Lo abbiamo dichiarato in tante situazioni e, recentemente, abbiamo visto quanto è successo sull'acqua pubblica e come il *referendum* sia stato straziato, ignorato e vilipeso. Noi crediamo si debba distinguere, invece, molto chiaramente tra mercato e volontariato, tra lucro e gratuità.

dei partiti, o di singoli esponenti di partiti o delle correnti interne. Quindi, per definizione, sono promotori di un interesse di parte (partito deriva proprio da parte) e pertanto non possono vedersi riconosciuta una finalità di natura sociale, universale, collettiva. Ricordiamo ancora che si tratta di associazioni ed enti in cui gli organi direttivi sono spesso occupati da o da esse nominati. Si tratta di società e associazioni che finanziano i partiti, direttamente e indirettamente, attraverso la fornitura di servizi, come studi e supporto logistico. Sono Sono enti finanziati, peraltro direttamente, da gruppi di interesse economico da *lobby*, come possono essere quelle dell'azzardo e del petrolio. Quindi, è troppo marcato il loro carattere di portatrici di interessi specifici per vedere loro riconosciuti benefici, sgravi e vantaggi di ogni natura che, invece, questa legge dovrebbe opportunamente riservare a chi persegue in modo gratuito un interesse collettivo. Sono almeno 60 le fondazioni di questo tipo censite nel 2015. La maggior parte di queste Grazie, si pronunciò in maniera molto pesante, dichiarando che si assisteva a una corruzione totale della vita politica e che l'attenzione doveva andare, non soltanto ai partiti o ai singoli esponenti, ma a questo sottobosco di organizzazioni dove manca la trasparenza. Bene, anche per questo motivo, in una legge delega andrebbe esplicitato tale principio. Non possiamo ammantare di finalità filantropiche organizzazioni che perseguono interessi a volte biechi e, in ogni caso, assolutamente particolari.

parliamo comunque di iniziativa economica privata in un ambito, quello della tutela dei diritti civili e sociali, che dovrebbe essere precipua competenza dello Stato, della Repubblica. Ora, non nego che l'iniziativa privata possa concorrere, ma che debba essere incentivata con risorse e benefici pubblici mi sembra discutibile. Proponiamo allora, con l'emendamento 2.204, di garantire e riconoscere il valore sociale dell'attività svolta gratuitamente, senza scopo di lucro diretto o indiretto, totale o parziale, e anche se questa svolta per la produzione di beni e servizi, che questo non sia in alcun modo veicolo di profitto, di lucro Questo è un principio che in una legge delega dovrebbe essere sottolineato, sottratto alla possibilità di equivoco ed all'eccesso di delega, che questo Governo ci ha abituati a vedere continuamente. Dobbiamo riprendere in mano il diritto del Parlamento di dare precise indicazioni prescrittive al Governo nel momento in cui delega la funzione legislativa.

tendono a dare una maggiore concretezza e precisione alla lettera *c)* del comma di cui stiamo parlando, che «assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti». Ora, rispetto alla dicitura «interessi coinvolti», potrebbero non essere quelli degli enti, ma, a parte questa indeterminatezza, noi dobbiamo capire di quale finalità stiamo parlando e dobbiamo inserire criteri prescrittivi al Governo per i futuri decreti legislativi. Poniamo quindi alcune indicazioni: per esempio, che si tratti di finalità solidaristiche, di tutela di interessi delle comunità a cui si rivolgono e ancora - e rispetto a questo veramente non capisco

Io credo che non possiamo enunciarli in maniera così astratta e vaga, come è nel testo che ci è giunto dalla Commissione (non per colpa della Commissione, ovviamente, ma perché queste erano le indicazioni evidentemente di una maggioranza

ribadisco la necessità di prevedere espressamente l'assenza di scopo di lucro, perché, se in una legge delega non la escludiamo espressamente, ciò vuol dire autorizzare il Governo ad introdurla. E, nel momento in cui autorizziamo il lucro nella gestione di servizi e di attività a scopo sociale, stiamo compiendo un misfatto che offende la Costituzione, che della solidarietà, della volontà, della gratuità, della reciproca collaborazione tra i cittadini e le forze sociali ha fatto un pilastro della nostra convivenza sociale. Stiamo autorizzando un misfatto; vi chiedo di escludere esplicitamente questa possibilità.

lo faccio qui, nel tempo che lei mi concede. Noi dobbiamo «prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del terzo settore qualora esercitata con finanziamento pubblico o per l'espletamento di servizi pubblici, non comporti maggiori costi o minore livello di prestazioni rispetto ai servizi pubblici presenti o attivabili dalle pubbliche amministrazioni includendo nei costi eventuali finanziamenti pubblici, erogazioni liberali,» - che sono sempre soldi dei cittadini - «raccolte di fondi comunque realizzate (...)». Ecco, io credo che questo sia un principio elementare, che andrebbe inserito. Noi abbiamo bisogno di verificare quale sarà l'impatto di questa normativa sul nostro sistema di *welfare*, altrimenti potremmo trovarci troppo tardi a scoprire che siamo stati scippati avendo indebolito quello che per il

mi devo rassegnare, almeno dal punto di vista delle dinamiche d'Aula (non in cuor mio, ovviamente), al fatto che non si vuole escludere l'iniziativa privata e il lucro. Però con questo emendamento si chiede almeno di subordinarlo nell'ordine delle priorità, e cioè di «promuovere i princìpi di solidarietà politica, economica» e a «valorizzare le attività improntate alla dimensione della gratuità rispetto a quelle di natura imprenditoriale». Vogliamo riconoscere almeno che non stanno sullo stesso piano? Questo si chiedo semplicemente.

«*al comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le parole*: "anche attraverso la pubblicazione nel suo sito Internet istituzionale"».

in quanto la questione è stata recepita e assorbita nell'emendamento del relatore 3.217, peraltro spostato nella lettera *a)* dello stesso comma 1.

debba essere prevista la pubblicità dei bilanci e degli emolumenti, dei compensi e dei corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Dobbiamo sapere quanto queste persone ricavano come retribuzione per la loro attività. Abbiamo visto come è possibile costruire degli imperi. Dobbiamo garantire l'assenza di conflitti di interesse. Sono norme che dovremmo inserire

Volpi, cerco di dare conto del nuovo testo Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale».

apra la strada per fusioni e trasformazioni tra associazioni e fondazioni, creando degli aggregati potenzialmente enormi, vere e proprie *holding* a volte. Questo in contrasto con il principio per il quale dovremmo valorizzare il contributo della pluralità delle voci, l'aderenza e il radicamento delle associazioni e degli enti sul proprio territorio. È un principio, peraltro, affermato anche nella Costituzione. Vorremmo sostituire questa lettera con una previsione, che prevede per il Governo, ad emanare una disciplina distinta per le associazioni e le fondazioni, articolandola in relazione agli interessi coinvolti, al patrimonio dell'ente, alla sua dimensione, ai rapporti interni e con i terzi. Dovremmo anche diversificare le situazioni in cui queste norme possono essere applicate anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. lo sforzo di differenziare, anziché favorire, come un effetto valanga, aggregazioni che poi portano ad enti più facilmente controllabili, magari sul piano della della gestione del consenso e dell'orientamento anche elettorale che ne può derivare, ma poi difficilmente ancorabili agli interessi delle comunità locali e ai fini che dovrebbero e dichiarano di voler perseguire.

sulla struttura organizzativa e sugli obblighi di trasparenza. Il Governo deve fare in modo che siano garantiti i requisiti di trasparenza, di informazione e di pubblicità. prevenire i comportamenti illeciti: abbiamo visto purtroppo, dolorosamente, anche qui a Roma, nel caso di mafia capitale, come ci possano essere degli inquinamenti. Non sto parlando delle associazioni di volontariato, ma di tutto ciò che può essere incluso, in maniera magmatica e indistinta, all'interno del provvedimento

l'articolo 4 disciplina i principi e i criteri direttivi a cui devono uniformarsi i decreti legislativi. Tale articolo è caratterizzato da enunciazioni

Signora Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 4 mirano ad ampliare e rendere più precisi i criteri di

Credo che su questo disegno di legge pesi un grande interrogativo e, cioè, se stiamo trasformando il volontariato in uno strumento per fare *business*,

Non è sufficiente dare una generica pubblicità dei contenuti degli statuti e delle linee generali. La pubblicità deve essere data per tutte le operazioni e le spese e deve essere obbligatoria non soltanto per quei

affinché questa legge possa, poi, essere monitorata dai cittadini stessi che dovrebbero essere fruitori, ma anche, in questo caso, animatori

il tema dei controlli è ampiamente trattato successivamente, all'articolo 7, e, per quanto riguarda la tutela del lavoro, ho già detto precedentemente.

Ciò è previsto, ma limitatamente ai volontari presenti negli enti di terzo settore. Quindi, per certi versi, la proposta recepita in Commissione e arrivata in Aula contiene

al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proseguendo poi come recita l'emendamento. Questo al fine di valorizzare il principio di proporzionalità tra i trattamenti economici, che in effetti era importante e che recepiamo esprimendo parere favorevole,

Grazie,

la possibilità per gli associati e i lavoratori degli enti del terzo settore di segnalare, all'interno dell'ente, eventuali illeciti e irregolarità secondo il modello del *whistleblowing*. Stiamo dicendo, cioè, che è interesse della categoria intera di questo settore, e delle tante realtà virtuose che veramente compongono una delle ossature di questo Paese, vedere tutelata la loro credibilità attraverso una più efficace possibilità di smascherare le poche realtà dove invece si perpetuano illeciti anche gravi, come abbiamo visto recentemente. Noi abbiamo bisogno di un'alleanza con tutti i soggetti che possono avere un punto di vista privilegiato, per far arrivare alla magistratura quanto prima ogni eventuale distorsione, a tutela di un patrimonio su cui si fonda la nostra convivenza.

si chiede di prevedere che gli enti del terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici nell'acquisto di beni e servizi rispondano ai parametri di prezzo e qualità fissati da Consip. Quando un ente del terzo settore procede ad un acquisto, utilizzando risorse pubbliche, deve anche essere vincolato ai criteri di efficace ed efficiente utilizzo di queste risorse. Proprio per il fatto che sta svolgendo in parte una funzione pubblica, deve sottostare agli stessi requisiti che l'attività amministrativa pubblica deve avere, cioè quelli dell'efficacia e dell'efficienza. Non possiamo permetterci che il fatto di beneficiare di finanziamenti pubblici consenta a questi enti ovviamente mi riferisco a quella piccola parte di situazioni dove si perpetuano degli illeciti o delle situazioni grigie - di garantire al venditore un lucro su materiali, beni o servizi offerti.

semplicemente il rispetto di una questione etica, e cioè che i componenti degli organi di amministrazione e controllo all'interno di questi enti non possono vedersi attribuiti compensi

realizzano attività e funzioni di solidarietà, di servizio, di tutela dei diritti civili e sociali, non ci debbano essere sperequazioni

con l'emendamento si chiede semplicemente di coinvolgere nei processi di valutazione anche i beneficiari delle attività e degli interventi. Laddove riconosciamo una funzione pubblica, in regime di sussidiarietà, a questi enti rispetto a compiti dell'amministrazione pubblica dello Stato, dovremmo

4.289 prevede che, laddove un ente del terzo settore svolga per oltre un anno attività esclusivamente e interamente per conto della pubblica amministrazione (risultando quindi implicitamente una sua emanazione o comunque avente un rapporto troppo privilegiato per essere considerato un ente totalmente svincolato), questo sia

che sia istituito un registro del terzo settore presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali. Noi riteniamo invece che tale registro debba essere costituito

in questo modo si sposti la funzione di controllo dal Governo, che in maniera troppo sospetta sta spingendo questo provvedimento con finalità che molto spesso non sono ben riconducibili a quelle dichiarate, e la si avvicini ai cittadini, a quegli organi pubblici che tutelano i cittadini e infine alle associazioni che

del terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Crediamo che ciò possa comportare il rischio di una riduzione della pluralità delle voci e, in qualche maniera,

processi aggregativi, che pure possono esserci, si debba garantire la rappresentatività presso i soggetti istituzionali anche degli enti minori - in qualche modo lasciamo al Governo la responsabilità di definirli, ma senza potersi

Penso - ad esempio - all'importanza che tante di queste realtà hanno a livello locale, dove spesso si realizzano la politica e l'amministrazione più virtuose e vicine ai cittadini.

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o

la giornata è iniziata dodici ore fa con i gravi attentati di Bruxelles. Non sfuggirà a nessuno che, mentre stiamo completando queste votazioni, le agenzie di stampa ci riportano gli eventi che sono sempre più

Governo. Abbiamo una preoccupazione che certamente il Parlamento deve dissipare con certezze che il Governo deve dare. Quello che sta accadendo ci scuote profondamente.

Presidente, visto il calendario dei lavori, i quali verosimilmente dovrebbero comunque concludersi domani, e visto che siamo oltre la metà nell'analisi dell'articolato, credo che potremmo interrompere qui e aggiornarci alla

Signora Presidente, intervengo a proposito della recente costituzione di un polo di ricerca di altissima qualificazione nell'area ex Expo.

Tale finanziamento è simile a quello dedicato dalla legge di stabilità, approvata qualche settimana prima, a tutte le settanta università italiane e ai dodici enti pubblici di ricerca.

grande polo di ricerca e in una conferenza stampa il Presidente del Consiglio annuncia il conferimento di ulteriori 150 milioni l'anno per dieci anni, pari a 1,5 miliardi di euro. di euro. Nei mesi fra novembre e febbraio il direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia ha effettuato quella che possiamo definire una operazione di *scouting*, cercando di coinvolgere, con metodi piuttosto oscuri e poco trasparenti, rettori di università pubbliche e presidenti di enti pubblici di ricerca, in particolare quello del CNR,

in quanto nega e confligge con una valutazione oggettiva, comparativa, trasparente e partecipata tra i possibili contenuti dello Human Technopole. Cari colleghi, signora Presidente, siamo in presenza di un vero e proprio cambiamento di rotta nella politica di ricerca di questo Paese. Siamo passati da una assegnazione delle risorse agli organismi pubblici sulla base di bandi competitivi all'erogazione di risorse a un ente privato che, con meccanismi oscuri, redistribuisce queste risorse ad amici e conoscenti. Preannuncio la presentazione di una interrogazione parlamentare per sapere chi e con quali modalità ha dato incarico all'Istituto italiano di tecnologia di procedere in questo modo, assolutamente deprecabile, per l'avanzamento delle conoscenze e la ricerca in questo Paese. *(Applausi

questo è quello che il Governo Renzi e la maggioranza PD, la sinistra italiana, stanno assicurando ai lavoratori. Mi riferisco in particolare al settore del lavoro stagionale,

persone a vivere oggi? Il Governo aveva detto, tramite qualche suo rappresentante, che avrebbe risolto il problema - abbiamo letto anche dichiarazioni rilasciate alla stampa - ma ovviamente, come sempre, sono soltanto balle.

della scuola. Erano ex LSU, persone che hanno sempre lavorato precariamente per lo Stato, e da questo trasformati in co.co.co e, quindi, in ulteriore precariato.

Signora Presidente, l'8 marzo, a Venezia, tra Italia e Francia, rappresentate rispettivamente da Matteo Renzi e Francois Hollande, è stato siglato il protocollo addizionale all'accordo del 24 febbraio 2015 inerente ai lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In merito a questo evento è stata diffusa una nota stampa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si evidenziano due punti principali: la validazione del costo certificato del progetto e criteri per la rivalutazione, e la questione dei controlli antimafia. Ora, è chiaro a tutti che, per quanto riguarda la questione della criminalità, il codice antimafia non si applicherà ai lavori TAV della Torino-Lione in territorio italiano, perché escluso dalla legge di ratifica (la n. 71 del 23 aprile 2014, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 7 maggio 2014) Grazie, non basta un impegno generico di lotta alla criminalità organizzata, che sembra essere presente nel nuovo accordo. Non basta neppure che il promotore TELT si doti di un proprio protocollo regolamentare sull'applicazione di codice antimafia, non avendo alcuna competenza legislativa. Necessariamente occorrerà usare lo strumento legislativo: occorrerà, quindi, un nuovo accordo tra Italia e Francia di abrogazione dei predetti articoli dell'accordo del 2012, da far poi confluire nel nostro ordinamento attraverso una nuova legge di ratifica. Questo è uno dei problemi, ma sicuramente ci sono altre opacità. Vorremmo anche approfondire - per esempio - la questione costo, ma è impossibile. È chiaro che la nota stampa della Presidenza del Consiglio non può essere considerata la base di lavoro di questa Camera né dell'intero Parlamento. Eppure, il testo dell'accordo, che deve essere ratificato in queste Aule, non è stato diffuso: è forse segreto? È forse questa la tanto decantata trasparenza del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro Delrio? Sollecito anche la Presidenza del Senato affinché si faccia carico della diffusione del testo firmato per permettere a tutti i senatori di averne contezza. Fino

sono solo fumo e niente arrosto, purtroppo. Tra l'altro, si tratta di un fumo acre, di bruciato. Forse sono i soldi dei cittadini italiani che vengono irrimediabilmente ridotti in cenere.